L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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 Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi

e di questo ringrazio tutti i componenti della Commissione e il rappresentante del Governo. Purtroppo, però, non è stato ancora possibile concludere il lavoro, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio che, a quanto ci risulta, tornerà a riunirsi domani mattina alle ore 9. Signor Presidente, chiedo dunque di rinviare l'esame del provvedimento

Signor Presidente, il disegno di legge n. 467 approvato dalla Camera dei deputati, con modificazioni di carattere formale, reca la conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, in merito al prolungamento delle operazioni elettorali. Il decreto consta di due articoli. L'articolo 1 autorizza il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023, che si terranno dunque, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche in quella di lunedì, limitatamente alla fascia oraria dalle ore 7 alle ore 15. Il comma 2, dell'articolo 1, quantifica in euro 14.874.000 euro i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta per l'anno 2023 e, pertanto, contempla un incremento dello stesso importo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e dell'attuazione dei *referendum*. In ragione di tale onere, il comma 3 dispone una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Il comma 4 prevede di conseguenza che il Ministro dell'economia e delle finanze possa apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 2 dispone inoltre l'entrata vigore del decreto-legge in questione.

tratta di una deroga - prevista per la corrente annualità - alla normativa vigente che prevede il voto nella sola giornata di domenica. Facciamo un breve *excursus*: breve *excursus*: fino al 1993 la normativa prevedeva che le operazioni di voto si svolgessero nell'intera giornata di domenica e nella giornata di lunedì fino alle ore La modifica che prevedeva le operazioni di voto nella sola giornata di domenica fu introdotta, appunto, con la riforma elettorale del 1993; quindi, le elezioni politiche del 1996 e del maggio 2001 si svolsero nella sola giornata di domenica. Nel 2002 si ripristinavano le operazioni di voto nelle due giornate, fino al 2013, con la legge n. 147, che ha ridotto a un solo giorno le operazioni di voto: la legge di stabilità per il 2014, appunto, nell'ambito di misure volte a conseguire risparmi di spesa. Quindi, la ragione che ha spinto a ridurre le operazioni di voto era ed è di carattere meramente economico e finanziario. Credo invece sia utile riconsiderare l'esito di questo risparmio, visti anche l'andamento delle ultime

Questa deroga è prevista solo per l'annualità 2023, quando si svolgeranno le diverse elezioni regionali che affronteremo,

da chi essere governati senza dover rinunciare a fare altre attività, ma potendo scegliere il momento più congruo ai propri impegni per esercitare il proprio diritto

il decreto-legge al nostro esame ha una sola previsione: poter fare votare gli elettori in due giorni, nell'anno in corso, come si faceva una volta, anziché in una sola giornata. È una disposizione che - come è stato detto - avviene in deroga alle norme della legge di stabilità per il 2014, momento dal quale si vota in un solo giorno. Ma se andiamo a vedere le percentuali delle elezioni degli ultimi trent'anni, notiamo che il calo di votanti c'è sempre stato. I votanti sono diminuiti sia quando si è votato in un giorno sia quando si è votato in un giorno e mezzo, posto che lunedì si vota fino alle ore 13. Nel 1992 alle elezioni politiche, con la legge proporzionale, i votanti sono stati oltre l'87

In queste tre tornate elettorali si è votato con la legge Mattarella, conosciuta anche come Mattarellum. Nelle tre tornate elettorali successive si è votato con la cosiddetta legge Calderoli, definita dal suo stesso creatore con il nome latinizzato di Porcellum, e gli elettori hanno sempre avuto a disposizione due giorni per esprimere il loro voto. Anche queste tre tornate hanno registrato un calo costante degli elettori.

La legge successiva, legge Rosato, nota anche come Rosatellum, è stata utilizzata, oltre che nelle elezioni anticipate del settembre 2022, anche nel 2018,

Possiamo notare che il calo dei votanti è stato lento e inesorabile. Che cosa hanno in comune queste leggi? Una progressiva riduzione della possibilità degli elettori di scegliere i propri rappresentanti; da una parte collegi uninominali, peraltro sempre più grandi, e - dall'altra - listini, in cui l'elettore può solo prendere o lasciare. In alcuni casi l'elettore lascia, alimentando ancora di più l'astensionismo. Dico questo conscia di essere stata io stessa eletta in un listino bloccato, di esserlo stata in quanto donna che seguiva un uomo che ha optato per un'altra carica elettiva incompatibile con quella di parlamentare. Non so quale sia la legge ideale per far tornare gli elettori alle urne, ma non sono nemmeno sicura che questa sia solo la causa, ovvero la concausa. Quello che appare evidente è che la legge elettorale, con una quota di maggioritario o di uninominale, funziona se gli schieramenti che si scontrano sono due. Ma, se l'elettore non si riconosce nei due schieramenti principali e nemmeno nel terzo o nel quarto polo, come è successo nelle ultime elezioni, tende a non andare a votare. la disaffezione alle urne è andata via via crescendo, e non solo per le elezioni politiche, ma anche per i *referendum* che - va ricordato - hanno prima di tutto il *quorum*, cioè il raggiungimento di almeno il 50 per cento degli elettori, per assegnarne la vittoria oppure la sconfitta. sconfitta. Personalmente conosco anche il vaglio delle preferenze, essendo già stata eletta all'Assemblea regionale siciliana, dove si ricevono i voti sulla propria persona da parte degli elettori, così come si ricevono i voti per essere eletti nei consigli comunali, dove vige ancora il sistema delle preferenze e dove si vota in due turni elettorali.

posto che diversi problemi che ho segnalato si riproporranno alle prossime elezioni regionali. Serve una classe dirigente politica credibile; servono programmi realizzabili; serve avere chiaro cosa si può promettere e cosa non si deve. È necessaria, cioè, un'ampia riflessione che porti a un salto di qualità della proposta della classe politica; altrimenti potremmo pure prevedere il voto in una settimana intera, ma il distacco degli elettori dalle urne sarà sempre più ampio, a marcare una sempre più larga distanza tra cittadini ed eletti.

tratta in modo chiaro ed esplicito del prolungamento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie per il 2023. Non può essere semplicemente un ragionamento economico e finanziario a limitare uno dei diritti più importanti, il diritto di voto, che è costituzionalmente garantito. un diritto personale, che non può quindi essere delegato. La Costituzione prevede anche che sia la legge a dover decidere le modalità e i requisiti con cui il diritto di voto deve essere esercitato:

Il voto non è un *optional,* anche se in Italia ci sono partiti che hanno governato per anni senza essere votati. E questa è la situazione più drammatica della democrazia. *(Applausi)*. Ricordo invece che maggiore è la partecipazione, maggiore è la democrazia e, di conseguenza, la legittimazione delle istituzioni agli occhi dei cittadini e degli elettori, così da ridurre quel distacco tra elettori ed eletti che sovente è proprio la causa della disaffezione.

Vorrei poi anche ricordare la problematica posta all'interno del dibattito sul voto dei fuorisede, che è un tema importante. Il primo a riconoscerlo è stato proprio il Governo, che in Commissione affari costituzionale e poi in Aula ha ribadito che sarà una priorità un dibattito franco, concreto e leale su come intervenire sul diritto di voto per i fuorisede, senza però ledere il principio democratico della rappresentanza.

né possiamo ignorare l'esercizio di un voto non orientato, quindi non cristallizzato in maniera perfettamente coerente e chiara, nonché il diritto dei territori ad esprimere la propria vocazione elettorale. Questo è un tema del quale bisogna parlare senza pregiudizi, con la consapevolezza che esiste una volontà politica che deve trovare la forma per potersi esplicare. Nessuno è in grado di governare un altro senza il suo consenso. Questo lo diceva Abraham Lincoln e credo che oggi tale affermazione sia più attuale che mai. Attraverso il consenso elettorale si attuano le scelte politiche di Governo, ma anche di rappresentanza, di maggioranza e di opposizione, in Parlamento, che determinano la reale portata e il valore di una democrazia, che per il nostro Paese ha un'importanza vitale, alla luce del fatto che proprio in questi giorni ricorderemo dei drammatici eventi della Prima e della Seconda guerra mondiale attraverso il Giorno della memoria. E questo ci riporterà indietro nel tempo,

La Presidenza del Consiglio scriveva una cosa e poi, all'atto pratico, ne faceva un'altra. Noi invece, con molta coerenza, teniamo fede a quel lavoro che era stato fatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e rendiamo operativo quello che ormai penso possano capire tutti: votando un giorno in più fino alle ore 15, ci sono buone possibilità che la gente vada più volentieri a votare e possa recuperare. Era giusto metterlo in evidenza, visto che

amministrative regionali e *referendum* che si svolgeranno nel 2023 possano svolgersi, oltre che la domenica, anche il lunedì fino alle ore 13. Siamo convinti della bontà di questa scelta, anche perché riteniamo che prolungare le operazioni di voto porti ad agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini, anche tenendo conto purtroppo del fattore crescente dell'astensionismo. Ricordiamo, infatti, che nelle ultime elezioni c'è stata una riduzione forte, significativa e importante dell'affluenza alle urne. Basti pensare

è un valore che non ha colori di appartenenza. Dobbiamo lavorare tutti affinché aumenti la partecipazione alle urne e, quindi, alla vita democratica della nostra Nazione, Il diritto di voto è uno dei diritti più importanti previsti dalla nostra Costituzione ed è una delle forme più significative di espressione democratica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, noi di Alleanza Verdi e Sinistra non ci opponiamo al disegno

il provvedimento in esame ha una finalità che tutti condividiamo: favorire la partecipazione elettorale dei cittadini in un'epoca di crescente astensionismo, esattamente come ci chiede di fare la nostra Costituzione. La partecipazione dei cittadini al voto è sicuramente garanzia di un rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni quanto abbiamo bisogno di rafforzare le istituzioni e il processo democratico, visto che negli ultimi vent'anni - come hanno sottolineato i colleghi - la partecipazione al voto è crollata di 20 punti percentuali:

In pratica in due decenni abbiamo perso più di 10 milioni di voti. Nelle elezioni di settembre i partecipanti sono scesi sotto i 30 milioni e le elezioni politiche sono le più sentite. Con il decreto-legge in esame si fa un piccolo passo in avanti, che certamente non sarà decisivo, ma darà comunque un contributo positivo. Il testo prevede di tornare a due giorni di votazione e questo sicuramente agevolerà la partecipazione - almeno ce lo auguriamo - anche in vista delle elezioni regionali del Lazio e della Lombardia. Quella che era una consolidata tradizione ha ceduto il passo agli interventi per ridurre la spesa pubblica e contenere il costo delle consultazioni elettorali. La riflessione che si impone oggi, però, è che il tema è troppo importante per essere ricondotto a una mera questione economica. Molto opportunamente nella passata legislatura il ministro D'Incà aveva affidato a una commissione di studio le ragioni della riduzione della partecipazione al voto; era stato redatto dal professor Bassanini un libro bianco che contiene una serie di proposte che meriterebbero di essere

Al tempo stesso sottolineiamo che all'interno del libro bianco ci sono alcuni suggerimenti che vanno oltre la data delle elezioni, la valutazione del progressivo invecchiamento della popolazione, con il risultato che molte persone anziane faticano a potersi recare al seggio per gravi difficoltà motorie. Di questo dovremmo tenere

La citata relazione della commissione di esperti ha quantificato in circa 5 milioni il numero di elettori che svolgono la propria attività lavorativa o studiano in luoghi diversi dal proprio Comune di residenza. Si tratta di circa il 10 per cento del corpo elettorale

per gli studenti e per i lavoratori fuori sede di votare dove lavorano e dove è il loro domicilio? c'è un ultimo aspetto che desidero segnalare, visto che affrontiamo questi argomenti, e riguarda la collocazione dei seggi elettorali. In Italia l'88 per cento dei seggi è all'interno dei plessi scolastici con l'ovvia conseguenza dell'interruzione temporanea delle elezioni. Anche su questo durante la pandemia abbiamo provato a ragionare: forse sarebbe arrivato il momento di collocare

Signor Presidente, voglio sgombrare subito il campo da possibili equivoci: il MoVimento 5 Stelle voterà favorevolmente questo provvedimento che prevede il prolungamento delle operazioni di voto alle prossime elezioni anche nella giornata del lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Dare più tempo agli elettori per recarsi alle urne significa favorire l'esercizio di questo diritto e tutti, specialmente qui dentro, sappiamo quanto sia importante, visti i tassi di astensionismo che purtroppo hanno caratterizzato le ultime tornate elettorali. Ogni strumento che sia in grado di aumentare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla vita politica e al voto in particolare è per noi il benvenuto. Per questo l'occasione ritengo sia quella giusta per ricordare a questa Assemblea che, oltre all'aspetto quantitativo del tempo per esprimere il voto, è necessario ampliare anche qualitativamente e metodologicamente gli spazi di partecipazione, includendo anche chi oggi è ingiustamente escluso o ha difficoltà spesso insormontabili per votare. Mi riferisco in particolare, naturalmente, ai fuori sede, soprattutto agli studenti, ai lavoratori, alle persone che sono lontane dalla propria città perché in cura altrove o perché accompagnano i propri cari a curarsi. Secondo l'Istat, nel nostro Paese si stima ci siano circa 5 milioni di persone alle quali viene sistematicamente preclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto. L'Italia è l'unico Paese in Europa a non permettere il voto a distanza a parte Malta e Cipro, che ovviamente per dimensioni hanno meno bisogno di una legge per il voto dei fuori sede. Negli ultimi quindici anni lo Stato ha investito oltre 60 milioni di euro per agevolare i viaggi di chi, appunto, si deve spostare per votare, ma questo si sta rivelando un sistema chiaramente inefficace e obsoleto. Vogliamo fare in modo che questa sia la volta buona e che in questa legislatura si possa finalmente superare questa stortura enorme che mina la democrazia nel suo cuore pulsante, cioè nell'esercizio del voto? Siete favorevoli - mi rivolgo, chiaramente, soprattutto ai colleghi della maggioranza - a istituire il certificato elettorale digitale o le innovazioni continuano a farvi paura, come avete dimostrato paventando addirittura di "spegnere" lo SPID? Se si vorrà intraprendere una strada di innovazione e di aumento della partecipazione, il MoVimento ci sarà, senza preclusioni ideologiche di nessun tipo. A fare le spese di questo *vulnus* tutto italiano sono, come dicevo, soprattutto i giovani, che per loro natura sono quelli che si muovono di più dalle proprie città e sono sempre più ai margini della vita politica. Ma come si possono prendere decisioni se di fatto i protagonisti delle conseguenze di quelle decisioni sono esclusi dal processo di partecipazione? A questo proposito, voglio anche ricordare che è soprattutto grazie all'impulso dato dal MoVimento 5 Stelle se nella scorsa tornata elettorale e per le future anche i diciottenni hanno votato per questa istituzione di cui facciamo parte, per il Senato. *(Applausi)*. Tutti noi, colleghi, colleghi, siamo qui anche grazie al loro voto ed è la prima volta nella storia della Repubblica italiana. Valutiamo, quindi, insieme se non sia il caso di fare ancora un passo in più e coinvolgere nel diritto di voto anche i sedicenni e fare veramente, concretamente, nei fatti, dei giovani uno dei pilastri su cui si fonda la partecipazione democratica per il futuro del nostro Paese, perché il futuro è il loro, così come questo Paese appartiene a loro. Presidente, colleghi e colleghe, non limitiamo lo sguardo ogni volta solo alla prossima tornata elettorale, proviamo ad alzare lo sguardo, proviamo ad esprimere una visione di Paese e di democrazia, cerchiamo di superare le ideologie e fare un percorso condiviso per ampliare la partecipazione. Questo decreto lo voteremo, come ho detto, ma facciamo in modo che sia l'occasione per far fare all'Italia quei passi avanti che un grande Paese come l'Italia merita. Il MoVimento 5 Stelle su questo fronte c'è. voi, colleghi della maggioranza, mi chiedo e vi chiedo, sperando che la risposta sia positiva, sarete in grado di dare una risposta a queste esigenze e di intraprendere un cammino verso più democrazia e più solida democrazia? *(Applausi)*.

il provvedimento che ci accingiamo votare è di buon senso e va incontro al diritto di voto che la nostra Costituzione sancisce nell'articolo 48. Purtroppo, limitare questo diritto a una sola giornata, quando gli impegni personali, familiari, lavorativi ci portano ad occupare anche la domenica, è sicuramente anacronistico. Questa proposta di legge, votata all'unanimità in Commissione, è un primo passo importante per l'appuntamento elettorale delle elezioni regionali nell'anno corrente. Tuttavia, è necessario considerare urgentemente di aggiornare la legge sulle operazioni di votazione per tre motivi: per questioni anacronistiche, come dicevo prima; per permettere a più persone di esercitare il diritto di voto; ma anche per migliorare la disaffezione alle urne, che in questi anni, appunto, è aumentata sempre di più, facilitando la volontà di andare a votare. Aggiungo anche che ormai è anacronistico utilizzare le scuole come sedi di seggi elettorali. Ormai gli appuntamenti non sono più saltuari. Tra scadenze di mandati

votare. Il nostro voto è sicuramente favorevole su questo provvedimento, ma per la partecipazione democratica al voto di tutti i cittadini, è bene andare a rivedere tutta la normativa sulle operazioni di voto per tutti gli appuntamenti elettorali.

perché sappiamo bene che una democrazia alla quale i cittadini non partecipano è una democrazia debole; e una democrazia debole è una democrazia incapace di svolgere quella fondamentale funzione di governo dei processi economici e sociali. Noi, però, vorremmo che quest'Aula, con la stessa condivisione con la quale si accinge a votare questo provvedimento, si esprimesse anche su alcuni disegni di legge che sono già incardinati in Commissione e sui quali è già persino stata svolta la relazione da parte dei relatori. Penso, ad esempio, al provvedimento che la scorsa legislatura, purtroppo, non è potuto giungere in quest'Aula, pur essendo stato approvato alla Camera, per garantire ai cosiddetti cittadini fuori sede circa cinque milioni di elettori - di esercitare il loro fondamentale diritto di voto. Abbiamo inoltre riproposto in questa legislatura, anche in quest'Aula, un disegno di legge che fa tesoro di quello che è stato il lavoro svolto da una commissione di esperti su come contrastare l'astensionismo involontario. preso spunto dai suggerimenti avanzati dagli esperti e abbiamo quindi ipotizzato una misura per garantire ai fuori sede, per ragioni specifiche e giustificate (lavoro, malattia, studio), di poter esercitare il diritto di voto attraverso l'istituto del cosiddetto voto presidiato anticipato. Questo disegno di legge è in Commissione e spero che venga rapidamente portato in Aula e approvato. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda disegno di legge che abbiamo presentato, volto a dare una più completa e organica attuazione all'articolo 49 della Costituzione. È difficile prendere sul serio il problema dell'astensionismo e quindi il problema della partecipazione alla vita democratica senza affrontare il problema di come far sì che i soggetti collettivi che organizzano la partecipazione e che rendono possibili i diritti politici tutti i giorni, e non soltanto al momento delle elezioni, siano messi in grado di svolgere questa fondamentale e insostituibile funzione. Abbiamo infatti presentato un disegno di legge, anche questo già incardinato e sul quale il relatore De Priamo ha già svolto la relazione, per

attuare concretamente il fondamentale diritto di prendere parte alla determinazione dell'indirizzo politico. Come ho detto all'inizio, noi voteremo a favore di questo provvedimento. Voteremo a favore dell'estensione, per le elezioni del 2023, Ma vorremmo che questo voto segnasse l'inizio di una seria discussione, che alla fine conduca all'approvazione di leggi da troppo tempo attese, per assicurare alla nostra democrazia quella legittimazione, quella solidità e quel riconoscimento che sono il presupposto indispensabile per conferirle la forza necessaria perché essa possa mantenere le promesse dell'uguaglianza e dell'emancipazione. Solo una democrazia davvero rappresentativa, solo una democrazia davvero partecipata può svolgere quella funzione emancipante che la nostra Costituzione le assegna.

deve saper fare autocritica e deve trovare i modi per coinvolgere e motivare maggiormente i cittadini. È pur vero che in tutte le democrazie mature il numero degli elettori è andato scemando, però a volte, quando le elezioni hanno la partecipazione è cresciuta. Penso agli Stati Uniti, una delle patrie della democrazia, dove abbiamo avuto elezioni importanti con percentuali elettorali più contenute e dove a volte i confronti politici più incerti e più accesi hanno fatto lievitare la quantità dei quantità dei votanti. Non c'è dubbio quindi che la politica deve saper avanzare proposte e proporre soluzioni che siano di interesse dei cittadini. Non è soltanto la durata dell'apertura dei seggi che determina la qualità della democrazia. Tuttavia noi siamo stati abituati per lungo tempo alla modalità elettorale della domenica e della seconda giornata del lunedì; ricordo, da giovane scrutatore o da elettore, che così sempre Poi si è deciso, in varie fasi, per ragioni di costi e di varia natura, di comprimere la durata del voto. Riteniamo che abbia fatto bene il nuovo Governo a ripristinare un arco temporale più ampio. non è nemmeno dettato da ragioni stagionali, perché questo turno elettorale si svolge in pieno inverno, in questi giorni di clima rigido e di neve, e altre volte si è votato in estate. Quindi i turni elettorali, che generalmente si svolgevano in primavera, ora stanno diventando un'eccezione, perché a causa del Covid abbiamo spostato dei turni elettorali a settembre e le stesse elezioni politiche - ma lì è stato frutto della crisi di Governo - si sono svolte per la prima volta a settembre. Quindi credo che ripristinare un arco di partecipazione più ampio per gli elettori sia un motivo valido per agire con il decreto-legge in esame e per agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini: non sto qui a dilungarmi sulle percentuali. Dopodiché non si deve ritenere - concludo con questo aspetto - che la qualità della politica e la partecipazione alla stessa si risolvano e migliorino solo perché oltre al voto della domenica abbiamo aggiunto alcune ore del lunedì. La capacità di coinvolgere i cittadini ricade su tutti noi, sulla serietà del nostro impegno, sulla coerenza del nostro agire e sulla reputazione della politica, anche cercando di far capire ai cittadini - non voglio polemizzare con nessuno - che in questo periodo si è potuto sperimentare di tutto. Nelle ultime legislature abbiamo avuto Governi di varia natura e abbiamo avuto Governi guidati da persone che non erano state nemmeno candidate alle elezioni. Dunque la democrazia ha determinato una possibilità ampia di scelta e allora, forse, i cittadini oggi devono sì fustigare i difetti della politica e criticare i partiti, ma anche riflettere su tante scelte che sono state fatte: forse non è vero che uno vale uno, non è vero che tutti quelli che proponevano i miracoli in terra poi li potevano realmente realizzare. Qui entrerei però in considerazioni di natura politica, che poco attengono al voto su un decreto-legge che si limita a determinare una diversa scansione temporale del turno elettorale del 12, ma anche del 13 febbraio. voglio infine cogliere questa occasione per ricordare a molti elettori che si vota: lei è lombardo e nella sua Regione si vota, io sono romano e nella mia Regione si vota. Pur partecipando, compatibilmente con i nostri impegni parlamentari e istituzionali, alla campagna elettorale,

spero che chi va a votare voti per il mio movimento politico, ma faccio un appello alla democrazia e alla partecipazione, quali che siano le scelte degli elettori, perché la libertà è partecipazione, come diceva una bella canzone di un grande protagonista della vita culturale del nostro tempo: Giorgio Gaber (come mi ricorda il senatore Speranzon, ma lo ricordavo anch'io). Vogliamo dunque che la gente possa partecipare e possa votare, perché la vera libertà

Signor Presidente, il provvedimento in esame, come illustrato compiutamente dal relatore, dispone la deroga alla normativa vigente in materia di operazioni elettorali e referendarie per l'anno 2023, quindi a cominciare dalle imminenti elezioni regionali del Lazio e della Lombardia, alle quali poi seguiranno quelle del Molise, del Friuli-Venezia Giulia e le elezioni amministrative per tutto l'anno in corso. Si tratta quindi di un provvedimento che al momento ha una validità annuale, ma per il quale ringraziamo il Governo, perché di fatto lo ha licenziato in tempi rapidi, per consentire di attuarlo fin dalle elezioni che si andranno a svolgere Si torna, almeno in questa circostanza, al voto in due giorni, così come è avvenuto fino al 1993 e come non è avvenuto dal 1993 fino al 2001.

dicevo, ha una validità limitata nel tempo, ma è certamente l'occasione per una riflessione sull'opportunità di una riproposizione anche in forma stabile del voto in due giorni: garanzia di una migliore attuazione del principio costituzionale relativo all'esercizio del diritto di voto. Negli ultimi anni, infatti, questo diritto si è progressivamente compresso, nel senso che è aumentata esponenzialmente la percentuale degli astenuti. Ovviamente non pensiamo che con una mezza giornata in più ci sia un cambiamento radicale, però, consentire di avere più tempo per recarsi alle urne significa maggiore partecipazione e quindi più rappresentatività per gli eletti.

ma sicuramente è un elemento importante. Nei Paesi anglosassoni, ad esempio, si vota durante la settimana lavorativa e c'è una percentuale sensibilmente più alta di votanti. In questo senso l'estensione al lunedì potrà dare un suo contributo. Ripeto, quindi, che sarà necessario riflettere e valutare l'opportunità di estendere le misure di questo provvedimento anche oltre

il Governo si porrà il tema e interverrà in modo adeguato. Tuttavia, in questi giorni di inizio legislatura ci sono altri temi che stiamo inserendo nella discussione per aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica. al ritorno del voto diretto per l'elezione dei Presidenti e dei consiglieri delle Province e delle Città metropolitane. Su questo vi sono disegni di legge di Fratelli d'Italia e di altri partiti della maggioranza, e andremo avanti con buona pace della sinistra, che ha votato la legge Delrio, motivandola con la volontà di eliminare le Province, quando, invece, le ha mantenute, privando, però, i cittadini del diritto di scegliere e di partecipare attivamente alla vita democratica di quegli enti. *(Applausi)*. A proposito di incentivi alla partecipazione, vogliamo anche mettere in discussione il dogma del doppio turno alle elezioni comunali, che troppo spesso ha fatto eleggere sindaci troppo poco rappresentativi. Insomma, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo provvedimento, riteniamo che sia un importante segnale, che sarà seguito da altri interventi verso un ritorno alla piena sovranità dei cittadini, dopo anni di disaffezione e di provvedimenti limitativi del diritto di voto degli stessi. La democrazia, infatti, perisce non solo quando viene sostituita, come, purtroppo, avviene ancora oggi in molte parti del mondo, dalle autocrazie o addirittura dalle dittature, ma anche quando di fatto diventa oligarchia, governo di pochi, perché, con motivi magari di copertura economica, vengono allontanati i cittadini dall'esercizio del voto. È avvenuto fino ad oggi, non accadrà più, perché vi è finalmente un Governo scelto dai cittadini e consapevole di quanto sia importante avvicinare e non allontanare i cittadini dall'esercizio del loro diritto di voto e dalla possibilità di scegliere da chi essere rappresentati.

Domani saranno quaranta anni che Cosa nostra uccise il magistrato Gian Giacomo Ciaccio Montalto nel territorio per troppi anni controllato da Messina Denaro. Due persone diverse, due tragici destini comuni. L'impegno di Guido Rossa era nel sindacato di Lama, nel partito di Berlinguer, nella fabbrica per i diritti del lavoro e dei lavoratori. Quando scoprì che nella sua Italsider si erano infiltrati cercavano di radicarsi brigatisti, terroristi che volevano colpire la democrazia, i sindacati, i partiti democratici e le stesse lotte operaie, Guido Rossa non ebbe paura, fece il suo dovere, denunciò responsabilità e connivenze, con grande coraggio e, in quel momento, anche senza troppa solidarietà. Averlo fatto gli costò la vita, ma il suo esempio ha rappresentato un contributo decisivo per far capire quanto le brigate rosse e il terrorismo fossero nemici del Movimento operaio e contribuì a isolarle e sconfiggerle. Nel ricordare Guido Rossa, vogliamo mandare anche un abbraccio

Liliana Segre, in una bella lettera, ricordando il sacrificio di Rossa e i suoi imponenti funerali, ai quali partecipò il presidente Pertini, afferma che il fatto che questo ricordo venga a ridosso del giorno della memoria non fa che rafforzare un bene prezioso perché la nostra società possa essere ogni giorno più libera dalla violenza e dal bisogno. Presidente, Gian Giacomo Ciaccio Montalto era un magistrato coraggioso che dopo aver indagato sullo scandalo petroli negli anni Settanta si occupò del contrasto alle mafie, al narcotraffico e al traffico delle armi. Per questo fu ucciso quella sera a Valderice, quel 25 gennaio. La figlia Maria Irene, qualche giorno fa ha detto che vorrebbe incontrare Messina Denaro per capire e chiedergli come sono andate le cose quel 25 gennaio, intendendo l'impegno dello Stato a ricomporre contesti, pezzi di verità e rapporti tra mafia e altri poteri.

che non si allentino strumenti di prevenzione e contrasto, comprendendo tra questi anche quelli di crescita culturale, intesa come cultura della legalità, crescita sociale e lotta alla povertà. Ecco, ci sentivamo di dire in questa giornata queste cose, in quest'Aula, nel ricordo di due persone per bene, due italiani come Guido Rossa e Gian Giacomo Ciaccio Montalto.

Signor Presidente, voglio unirmi al ricordo che il senatore Verini ha appena fatto rispetto all'uccisione di Guido Rossa, avvenuta il 24 gennaio 1979. Voglio anche dire con grande nettezza che la città di Genova pagò un prezzo altissimo proprio in riferimento alle

Presidente, non stiamo parlando di argomenti banali, ma di argomenti molto importanti per la vita del nostro Paese.

Mi faccia dire che, in virtù di questo ricordo e anche del prezzo altissimo che il nostro Paese ha

tutti ricordati e tutti citati anche in un'attività di indagine delle nostre Commissioni. Lo dico in quest'Aula nel ricordo di Guido Rossa, perché non ci sia differenza tra una morte e l'altra e perché il nostro Paese possa fare chiarezza indistintamente su *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo i miei natali a una città lucana meravigliosa, situata in provincia di Potenza, Muro Lucano, medaglia d'oro al merito civile. un territorio denso di arte e cultura, che affonda le proprie radici in millenni di storia. Basti pensare alla celebre località Raia San Basilio, che fu teatro di uno scontro fra Annibale e Marcello nel 210 Qui nei secoli si sono stratificate diverse culture e popolazioni che hanno lasciato traccia di sé, impreziosendo la nostra storiografia di reperti dal pregiato valore archeologico. questo la creazione di un museo archeologico nazionale è stata la risposta più ovvia all'esigenza di un territorio che reclamava a gran voce un luogo dove poter sfogliare i capitoli più significativi della propria esistenza. Non fu scelto un luogo qualsiasi, bensì il cinquecentesco seminario vescovile della città, che accoglie da anni numerosi reperti catalogati, preservati e restaurati. In questo sito d'interesse nazionale, ad esempio, è possibile ammirare la ricostruzione di un settore della necropoli arcaica dell'insediamento di Baragiano, in cui sono stati riposti i più significativi corredi funerari, così come i reperti rinvenuti nel centro antico di Raia San Basilio e presso il santuario ellenistico di contrada Fontana Bona di Ruoti. sono solo alcuni esempi dei beni più preziosi che annualmente migliaia di turisti, tra cui numerosi istituti scolastici, ammirano presso questo centro di eccellenza. punto, però, è un altro. Infatti, se da un lato è un onore illustrare nella sacralità di quest'Aula l'elevato pregio del museo, dall'altro è un onere lanciare un appello al Ministero della cultura. Purtroppo porto all'attenzione del Governo il grido d'allarme lanciato dal sindaco di Muro Lucano e da molti colleghi dell'area interessata, secondo cui il museo rischierebbe di chiudere alla luce dell'esiguità del personale e della prossima quiescenza di alcuni lavoratori. Perciò, alla denuncia che porto quest'oggi in Aula, seguirà una mia interrogazione parlamentare in cui chiederò al Ministero della cultura quali iniziative intenda intraprendere al fine di tutelare il museo e se condivida l'opportunità di sostenere l'assunzione di nuove unità lavorative. Al di là di ogni colore politico, l'auspicio è che il Governo dia rispose rapide e immediate, perché la cultura non deve essere perimetrata all'interno di steccati partitici.

si unisce ai sentimenti espressi in ricordo di queste due figure: Giacomo Ciaccio Montalto e Guido Rossa. Guido Rossa fu un sindacalista, iscritto alla CGIL e al Partito Comunista Italiano, che ebbe il coraggio di opporsi, proprio nell'ambito di quello

vicinanza da parte di frange della sinistra non violenta, per cui le brigate erano definite le brigate cosiddette rosse, compagni che sbagliano e così via. L'impegno di Guido Rossa - non lo chiamo sacrificio perché naturalmente avrebbe ben preferito non andare incontro a questa sorte - ha avuto il merito intanto di essersi opposto al fatto di portare avanti idee violente e il merito di aver segnato con quel suo straordinario atto atto la fine di quel periodo; da quel momento in poi, ogni vicinanza verso le brigate rosse da parte di qualcuno che poteva, in qualche modo, forse lontanamente, forse sotterraneamente condividerne alcuni aspetti, è finito. Per questo merita una commemorazione. Ricordare quegli anni non è sbagliato, perché sono stati anni difficili e di violenza politica; come ha detto la collega Paita, tutte le vittime vanno ricordate, in particolare chi ha compiuto atti particolarmente onorevoli e valorosi. Dobbiamo fare di tutto perché momenti come quello non tornino, e conoscere meglio quei fatti credo che sia un aiuto in questo senso.

la validità e l'esempio delle figure che sono state citate, ma anche per sottolineare che in quest'Aula tutto possiamo fare tranne che riscrivere la storia.

nei confronti delle brigate rosse cominciò con la morte di Guido Rossa è un falso storico, non è vero, non è la verità. *(Applausi)*. Fu ben altra la storia degli anni fu ben altro il lavoro politico che fu fatto in particolare dai militanti, dalle donne, dagli uomini, dai giovani del Partito Comunista Italiano, della FIGC, ma anche di tanti settori della stessa sinistra extraparlamentare che, pur mettendo in campo spesso politiche radicali, non condivisero per nulla la deriva armata di alcuni gruppi, ne contestarono radicalmente la modalità e non soltanto ne

Questo non è cominciato quando è stato ammazzato Guido Rossa, ma molto prima ed ha attraversato la storia e il sangue di uomini e donne che ci hanno appunto rimesso la vita, come nel caso di Rossa, o come tutti quei dirigenti e quei militanti comunisti e della sinistra che, anche a prezzo di scelte e sacrifici molto duri, combatterono la deriva terrorista nei luoghi in cui erano: nelle scuole, nelle università, nelle fabbriche. Non si falsifichi la storia, perché non facciamo un buon uso della storia stessa. Penso che su questo abbiamo invece il dovere di ricordare le cose come andarono.

una volta di più tutti gli esponenti della magistratura, delle Forze dell'ordine, cittadini comuni e persone del mondo del lavoro che sono state vittime del terrorismo politico

Non sarei intervenuto e lo faccio, pur senza intenti polemici (il Parlamento è anche un luogo di riflessione politica), dopo aver sentito alcune considerazioni del senatore De Cristofaro. Io non voglio datare datare fenomeni che sono stati diversamente valutati, però voglio ricordare a me stesso, per la mia esperienza di militante politico e anche di giornalista, anche perché gli anni mi consentono di averne memoria diretta, che non fu facile la maturazione di alcuni giudizi nei confronti delle brigate rosse. Io ricordo che una terribile strage fatta non dalle brigate rosse, ma da Potere operaio a Roma a Primavalle, quella in cui morirono i fratelli Mattei nell'aprile del 1973, a lungo fu considerata una faida interna di missini *(Applausi)*. Lo dico al senatore De Cristofaro: non lo dicevano dei militanti avversi, lo scriveva il giornale più venduto della capitale, che oggi rispetto ed è un'altra storia; quindi non sto chiamando in causa

prima uccisione politica, il primo omicidio delle brigate rosse (che non è stato ricordato nemmeno nella recente *fiction*, ben fatta e molto bella su Dalla Chiesa), a via degli Zabarella a Padova, quando furono uccisi Mazzola e Giralucci,

del programma, però furono uccisi. Per molte settimane si disse che anche quella era una faida interna di non si sa chi. «L'Unità» per molti anni pubblicava

Posso parlare? Hanno parlato altri colleghi, non sto offendendo nessuno. Giorgio Bocca, personaggio importante nella storia del giornalismo italiano, per molto tempo ha scritto articoli di un certo tipo; non voglio parlare dei manifesti contro il commissario Calabresi, sottoscritti da fior di giornalisti. Ce ne sono alcuni che vanno ancora oggi in televisione tutti i giorni, ma sottoscrissero il manifesto di vituperio - e uso un termine ottimistico - del commissario Calabresi, che poi fu ucciso e decenni dopo è stato condannato Sofri. È chiaro che poi la sinistra ha pagato un prezzo, quando nelle fabbriche la lotta all'infiltrazione terroristica è stata fatta da eroici sindacalisti, come Guido Rossa, o quando nella Fiat furono licenziati i famosi 41 sospettati. Ci sono state pagine di coraggio: ricordo anche la figlia di Guido Rossa, che è stata eletta poi in Parlamento anni fa. Nessuno vuole minimizzare la storia, però c'è stata,

sedicenti brigate rosse che erano nere. Quindi, è chiaro che la critica da sinistra al terrorismo c'era stata, ma all'inizio ci fu un po' di fatica a farla. *(Applausi)*.